Oscar Mammì, repubblicano, deputato per sei legislature, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, anche attore: un uomo garbato, disponibile al dialogo, capace, nei suoi quattro anni di incarico di Ministro, di legare il suo nome alla prima legge organica sull'emittenza radiotelevisiva. Non era facile in quel periodo tant'è che, all'esito favorevole del voto del Parlamento alla sua riforma, si dimisero dal Governo Andreotti ben cinque Ministri della sinistra democristiana. Ma non era facile soprattutto perché fu la prima legge organica di riordino del settore televisivo dopo quindici anni di non regolamentazione, o meglio, come qualcuno allora disse, di caos delle frequenze. Dico queste cose con radicato convincimento perché in quegli anni fu uno di coloro che attendevano con ansia una legge che desse certezza a un settore in rapida e incredibile espansione, ma che pagava fino in fondo la mancanza di punti di riferimento normativi che potessero guidare i tanti investimenti in un mondo che, a al di là dei contorcimenti, delle polemiche e dei demagogismi, ha sicuramente portato più libertà al nostro Paese. Da giovane liberale qual ero allora, ho sempre guardato al Partito Repubblicano come ad una sorta di partito fratello, con cui si hanno solide radici comuni (l'amore per la libertà e per il progresso, l'orrore per ogni dittatura, il rigido rispetto delle regole democratiche), anche se poi le singole scelte ci hanno diviso. In particolare, del Mammì repubblicano ho sempre rispettato e ammirato la grande capacità di dialogo, il valore che dava al riformismo, il fatto di riuscire a trovare sempre un compromesso nobile, che non fosse al ribasso e che rispettasse le convinzioni di tutte le parti. Ero direttamente interessato, quindi, a quello che stava succedendo nel panorama dell'emittenza televisiva e avevo vissuto in prima persona le battaglie per arrivare, anche in Italia, a un'autentica libertà di espressione: battaglie dure, fatte di accensioni notturne di ripetitori formalmente fuori legge e di trasmissioni semiclandestine, pagate spesso con provvedimenti di chiusura di radio e TV e di condanne nei tribunali. Sento spesso dire - l'ho letto anche su vari quotidiani in questi giorni - che la legge Mammì si è limitata a prendere atto dell'esistente; non è così o, meglio, non è stato solo così. Certamente il ministro Mammì intese confermare con il suo testo le conquiste di libertà che le televisioni e le radio private, nazionali e locali, avevano ottenuto sul campo. E già per questo gli dobbiamo essere riconoscenti, perché lo fece malgrado l'opposizione durissima di tutto il Partito Comunista e di parte della Democrazia Cristiana, allora partito di maggioranza; all'approvazione della legge con la fiducia, posta dal presidente del Consiglio di allora Andreotti, si dimisero - come ricordavo in premessa - ben cinque Ministri della sinistra democristiana. Ripeto, non si trattava solo di una fotografia dell'esistente, ma di una legge che per la prima volta riusciva a mettere a sistema in modo organico l'intero mondo delle radio e delle tv private, che fino ad allora era cresciuto senza regole e, anzi, contro la legge anacronistica che regolava al tempo il settore. Affermava inoltre una serie di principi cardine, cui ancora oggi ci atteniamo: che il pluralismo dell'informazione si dovesse applicare anche in ambito radiofonico e televisivo, che una regolamentazione di radio e tv non potesse prescindere da una regolamentazione della pubblicità, che si dovesse tenere conto degli incroci proprietari con l'editoria tradizionale. Era una legge per certi versi coraggiosa, che fu approvata solo grazie alla determinazione di Bettino Craxi e soprattutto alle capacità di Oscar Mammì: le grandi abilità di mediatore, la gentile ostinazione di chi sa di essere nel giusto, la facoltà di riuscire a vedere ben oltre il contingente, privilegiando il bene del Paese rispetto agli interessi di parte. Presidente, nell'avviarmi alla conclusione voglio cogliere l'occasione per salutare la figlia Alessandra, che sta assistendo ai nostri lavori Infine, voglio ricordare la sua grande dignità nei momenti difficili (difficili per tutti allora, anche per il Partito Repubblicano), ai tempi di Tangentopoli, quando non volle partecipare alla sanguinosa resa dei conti di quegli anni, convinto della sua onestà e del primato della politica. Presentò le dimissioni dal Parlamento con discrezione, quasi in silenzio. Signor Presidente, oggi il Senato ricorda Oscar Mammì, un dirigente politico del Partito Repubblicano Italiano, a lungo parlamentare, più volte uomo di Governo. Si è spento nei giorni scorsi, dopo una malattia che ha reso difficili gli ultimi anni di una lunga vita, ricca di obiettivi raggiunti e molto ben spesa, sia nella dimensione privata che in quella pubblica, mai venendo meno ai legami della sua famiglia e mai abdicando alla sua grande passione per la politica. Ha vissuto circondato dall'amicizia e dalla simpatia di chi l'ha conosciuto, dalla stima dei colleghi parlamentari e dal grande rispetto di quanti hanno avuto l'onore di collaborare con lui. Le senatrici e i senatori del Partito Democratico sono particolarmente vicini alla famiglia di Oscar Mammì, ai figli e ai nipoti, ai quali esprimono il loro affetto, nel ricordo di un collega dal quale molti hanno imparato a fare politica. Rivolgo un mio pensiero particolare alla figlia Alessandra, che ci ascolta dalla tribuna, e alla quale mi lega un'amicizia antica e forte. Se debbo sintetizzare in una sola frase la personalità politica di Oscar Mammì, dico che è stato un grande democratico, un laico, saldo nel difendere l'appartenenza dell'Italia all'Occidente democratico, leale su una linea di centrosinistra sinceramente *liberal* nel sistema politico. Se debbo ricordare con altrettanta brevità il suo profilo più personale, lo ricordo come un amico allegro e ironico, un uomo colto e pieno di interessi, aperto al nuovo e nemico delle avventure. Sono, ovviamente, numerosissime le iniziative di Oscar Mammì da parlamentare e da Ministro, ma non credo che oggi, qui in Senato, elencarle tutte possa essere il modo giusto per onorarlo. Voglio solo soffermarmi - lo ha già fatto adesso il presidente Romani - sui difficili anni del suo lavoro di Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, quando la realtà delle cose mise l'Italia davanti alla necessità e all'urgenza di promuovere un riassetto profondo del sistema televisivo nazionale. Ricordo quel tempo è allora che Oscar Mammì si è trovato ad affrontare la questione più delicata, più controversa e più difficile di tutta la sua carriera politica. Aveva davanti un nodo che la politica che lo aveva preceduto aveva sempre scansato, secondo il metodo del rinvio che allora era così di moda e che negli anni è costato tanto all'Italia. Il groviglio era molto duro da sciogliere per le sue implicazioni di carattere economico (la televisione è una grande industria e occupa decine di migliaia di lavoratori), sociale (l'Italia politica

In più c'era la condizione di illegittimità in cui operava il principale operatore privato, che allora trasmetteva su tutto il territorio nazionale senza tener conto dei divieti di legge ma contando su un'assenza di controlli che finì solo per opera della magistratura. In questo quadro, il costume del tempo avrebbe suggerito di rinviare nuovamente il problema a tempi migliori. Oscar Mammì non si tirò indietro e cercò la soluzione che a lui sembrava migliore, considerando la televisione non un tassello del meccanismo del potere in Italia, quanto un servizio che lo Stato era tenuto a regolare nell'interesse dei cittadini. Trovò la soluzione in una legge che porta il suo nome e che, in sostanza, decretava la fine del monopolio della RAI, l'inizio del duopolio con Mediaset e la legalizzazione delle televisioni locali private. La legge Mammì determinò una grande apertura del mercato televisivo, ma provocò anche polemiche politiche, sfociate nelle dimissioni di diversi Ministri. Oggi sarebbe insensato tornare a discutere su chi allora aveva ragione e chi aveva torto, io stesso, oggi, non sono più certo delle mie opinioni di allora. Parliamo di quasi trent'anni fa e tutto è cambiato. In Italia, oltre alla RAI, abbiamo ben tre grandi compagnie televisive che coprono tutto il territorio nazionale e la concorrenza si è fatta durissima sia sull'*audience*, che sulla pubblicità. Voglio invece dire qualcosa sulla persona di Oscar Mammì e sulle condizioni nelle quali maturò la sua decisione di varare quella legge, anche sapendo, lui uomo di centrosinistra, che sarebbe stata proprio la sinistra che lo avrebbe attaccato e si sarebbe opposta con tutte le sue forze. Negli anni Cinquanta John Kennedy, allora senatore del Massachusetts, scrisse un libro sul coraggio politico, un libro con cui vinse il premio Pulitzer. Kennedy sosteneva questa tesi: un uomo politico mostra coraggio non quando si oppone agli avversari (perché è naturale che ci si opponga agli avversari politici), ma quando, per sostenere una tesi in cui crede e per fare quel che ritiene possa servire al suo Paese, affronta battaglie politiche anche dure contro il pensiero della sua stessa parte politica, rischiando l'isolamento, l'ostracismo e la condanna dei suoi stessi alleati. A me oggi, commemorando Oscar Mammì, non importa se la sua legge fosse allora la migliore possibile; importa invece sapere che Oscar Mammì pensava che quella legge servisse all'Italia averla, ha lottato persino con i colleghi della sua stessa parte politica. È per questa ragione che oggi possiamo dire che Oscar Mammì possedeva quella dote rara che è il coraggio politico. Dobbiamo meditare su questo punto, perché l'insegnamento di Mammì vale anche per noi. È facile - in Parlamento lo facciamo quotidianamente e lo abbiamo fatto anche stamattina - battersi e inveire l'uno contro l'altro, maggioranza contro opposizione, ma il coraggio politico, come abbiamo visto parlando di Oscar Mammì, è un'altra cosa. Signor Presidente, perché è impossibile parlare di Mammì senza ricordare che egli apparteneva all'illustre famiglia del Partito Repubblicano Italiano, insieme a Ugo e Giorgio La Malfa, Bruno Visentini, Giovanni Spadolini, Dodo Battaglia, Chinchino Compagna e tanti altri.

che senza la grande scuola dei piccoli e nobili partiti di Ugo La Malfa, Giuseppe Saragat e Giovanni Malagodi e il loro lavoro di ricucitura delle fratture del Paese, la democrazia e la Repubblica italiana non sarebbero mai uscite forti e vitali dal buio del Dopoguerra. Il Partito Repubblicano è stato una fucina e una fabbrica di dirigenti politici; nei tanti anni del Dopoguerra tutti i partiti lo sono stati, ma i repubblicani, pur numericamente così pochi, lo sono stati più degli altri. Oscar Mammì non è stato mai settario, né massimalista. Non è stato mai un demagogo, né un superficiale, né un moralista. Poteva permettersi coraggio politico perché veniva da quella scuola lì e perché da quella scuola aveva assimilato i principi dell'amor di Patria.

che lo ha ricordato insieme a Stefano Folli la scorsa settimana, non è mai stato senatore. Però dall'altro ramo del Parlamento e dal Governo è stato più che un protagonista dell'Italia repubblicana;

1968, ma già durante la Costituente egli era il segretario della Federazione giovanile del Partito Repubblicano Italiano. Per Mammì e per molti giovani e meno giovani di allora,

Per Mammì il Partito Repubblicano Italiano - anch'esso partito ideologico, come disse una volta - nasceva in un mondo lontano, eppure irrinunciabile: il mondo del Risorgimento, la Roma che il suo amico Spadolini gli diceva di evocare, la Roma di Ciceruacchio, la Roma di Angelo Brunetti, la Roma di un laicismo molto forte, alla ricerca però di una convivenza con la Roma di Pio IX, se volete con quella di Giulio Andreotti. Da questo punto di vista, Mammì è stato un grande maestro di convivenza liberale,

ma io evocherei soprattutto Oronzo Reale e quelle risorse di finezza intellettuale e di sdrammatizzazione di tutto con una battuta, che sono irrinunciabili nella democrazia parlamentare. Come ha ricordato con molto affetto Paolo Romani, Oscar Mammì si distaccò dalla politica con discrezione, con eleganza,

del principio degli anni Novanta. È un libro edito da un senatore, nostro collega per molte legislature, Stefano Passigli, che si avvale Grazie,

né Reale sarebbero mai approdati in Parlamento, ma soprattutto la lotta politica avrebbe avuto un'asprezza totalizzante e totalitaria.

l'assemblearismo e la tolleranza per le opinioni degli altri sono state un difetto? Oggi questo "gargarismo" contro la partitocrazia

nel suo distacco e nel suo buon umore: la famiglia, collega Zanda, ma anche gli amici, il gioco delle carte, lo sdrammatizzare tutto e tutti. Finché ha potuto lo ha fatto, poi tutto deve avere un limite: Mammì ci ha abbandonato e molti di noi, in quest'Aula e altrove, si sentono più soli. Da qui, signor Presidente, il cordoglio dei senatori del mio Gruppo e l'affetto che ci lega, in giornate come queste, ai suoi familiari.

quella che tutti ricordano come la certificazione del duopolio RAI-Fininvest, al centro di uno scontro politico fortissimo, che provocò le dimissioni dal Governo Andreotti, composto da esponenti di ben sei partiti, dei ministri della sinistra democristiana: Sergio Mattarella, Mino Martinazzoli, Carlo Fracanzani, Riccardo Misasi e Calogero Mannino, contrari al via libera al disegno di legge, visto come un regalo al gruppo Fininvest di proprietà di Silvio Berlusconi e anche all'apposizione della questione di fiducia. Mammì, romano, nato nel 1926, laureato in economia e commercio, aveva iniziato a lavorare in banca prima di approdare alla politica ed essere eletto in Parlamento nella fila del Partito Repubblicano Italiano di Ugo La Malfa nel 1968. Parlamento è rimasto fino al 1993. Sono anni in cui ha ricoperto importanti incarichi nel partito e nel Governo. Fu Ministro per i rapporti con il Parlamento dal 1983 al 1987 e Ministro delle poste dal 1987 al 1991: gli anni in cui fu posto il problema del nuovo assetto radiotelevisivo, che fu risolto con la fine del monopolio della RAI e la "legalizzazione" di Fininvest. Riuscì a condurre in porto una delle leggi più scottanti e complicate dell'ordinamento italiano, quella che avrebbe posto fine al cosiddetto *far west* dell'etere, esploso dopo la famosa sentenza n. 202 del 1976, che aveva sancito l'incostituzionalità del monopolio RAI in tema di diffusioni radiotelevisive. In realtà si trattò per gran parte di una legificazione, cioè di una presa d'atto dell'equilibrio consolidatosi a seguito di numerosi pronunciamenti della magistratura civile, penale, amministrativa e soprattutto costituzionale. Tra i più importanti risultati conseguiti dalla legge n. 223 del 1990 vi fu l'inibizione dell'attivazione selvaggia di frequenze, che proseguiva da almeno quindici anni, determinando una profonda instabilità nella gestione imprenditoriale delle emittenti radio-televisive. Per converso, la legge cristallizzò il sistema impedendo l'ingresso di nuovi operatori (che avrebbero potuto solo acquistare imprese esistenti), ma consentì finalmente l'interconnessione strutturale in ambito nazionale (fino a quel momento era possibile solo quella funzionale, con la cosiddetta cassettizzazione), aprendo così anche ai telegiornali privati. Ancora oggi, gran parte del testo unico della radiotelevisione si fonda sui capisaldi della legge Mammì. Nel 1993, Oscar Mammì si dimise dal Parlamento. Era il periodo di Tangentopoli, quando ci si dimetteva dal Governo per un avviso di garanzia anche quando c'era il solo sospetto che potesse arrivare (sembra un periodo lontanissimo). Questo Questo sospetto aleggiava su Mammì dopo l'arresto di Davide Giacalone, suo principale collaboratore nella stesura della legge sulle televisioni. Il clima era tanto avvelenato che lo stesso giornale del suo partito scrisse il giorno delle sue dimissioni: «Non siamo ipocriti e in queste ore misuriamo sulla nostra pelle la sferzata della vergogna». Vero è però che il buon Mammì aveva sempre avuto la schiena dritta e di questo bisogna dargli sicuramente atto. Una vergogna che alla fine travolse però tutto il Partito Repubblicano Italiano, distruggendo un capitale politico liberaldemocratico che era stato costruito intorno alle parole d'ordine di competenza ed onestà. Il parlamentare Mammì non partecipò ufficialmente alle complicate vicende delle scissioni del partito e della diaspora dei suoi dirigenti nel centrodestra

in questo ruolo dell'Innominato, disse: «Andreotti è perfetto. Perché incarna il vero potere, che può servire il male ma anche il bene». E ne ebbe anche per i leghisti: il ruolo dei «bravi» lo affibbiò a Bossi, Calderoli e Castelli. «Ma sono finti cattivi» - spiegò - «giocano a mostrare il coltello, ma non lo usano mai. Dei bravi per bene», era convinto, e ammise che «uno che fa politica o è un bravo attore o non ce la fa». E di conseguenza il ruolo di Pinocchio lo affidò a Silvio Berlusconi. Per D'Alema evocò il ruolo del Conte di Montecristo: «giusto *mix* di cinismo e lucidità». Un quadretto ironico e colto, condito da una palese nostalgia: «Io ho vissuto una grande stagione, quella dei partiti: oggi è la stagione dei personaggi». Riteneva che: «Il potere dopotutto è sempre quello. È cambiata certo, sicuramente in peggio, la nostra democrazia: un tempo si lavorava per costruire il consenso, ora si cerca di sapere dove va il vento e lo si segue». Poi il silenzio e una lunga malattia. E un libro sullo scopone, quel gioco di carte che amava

Oscar Mammì è stato Ministro per i rapporti con il Parlamento durante il più lungo Governo della Repubblica italiana guidato da Bettino Craxi, quando l'Italia è diventata la quinta potenza economica del mondo. Mammì riusciva a tenere i rapporti con il Parlamento in maniera mirabile e non dimentichiamo che,

quel Ministro per i rapporti con il Parlamento sono riusciti a far passare un decreto speciale emanato dall'allora presidente del Consiglio Bettino Craxi, che ha impedito di escludere tali

Grazie, sono dovuti passare sopra anche alle dimissioni di cinque Ministri dell'allora Governo di centrosinistra. Ricordo una mia visita ad Hammamet a Bettino Craxi durante la quale mi rammentò che il Partito Comunista, per nome e conto dell'allora suo suo capogruppo Gerardo Chiaromonte, diceva di votare no, ma non impediva che fosse approvata questa importante legge in quanto c'era la fiducia e l'allora giovane responsabile della comunicazione, Walter

dire che questi erano politici illuminati che hanno fatto grande l'Italia. È per questo che credo sia

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il 10 giugno scorso è mancato Oscar Mammì. Era nato a Roma nel 1926 e sin dal 1946, a vent'anni, aveva scelto di militare nelle file repubblicane, nel corso della campagna sul *referendum* istituzionale. Laureatosi in economia e commercio, aveva iniziato a lavorare al Banco di Napoli, rivestendo ruoli sindacali e continuando l'attività politica militante nelle file del partito dell'edera, che è stata, come per tanti della sua generazione, la sua grande scuola di formazione politica. Nel 1968 venne eletto per la prima volta in Parlamento, ove rimase sino al 1994, affiancando all'attività di deputato quella di membro del Governo, prima come Sottosegretario all'industria e al commercio e poi, durante gli anni Ottanta, nelle vesti di Ministro per i rapporti con il Parlamento nel primo e secondo Governo Craxi, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni nei Governi Goria e De Mita e nel sesto Governo Andreotti. Il suo nome è indissolubilmente quanto indebitamente legato alla cosiddetta legge Mammì sulla riforma del sistema radiotelevisivo, ma questo dato di fatto ha contribuito a oscurare il resto della sua lunga e qualificata attività legislativa, che vorrei qui riproporre almeno in un punto saliente. Anzitutto, come Presidente della Commissione interni svolse un ruolo di grande mediatore che portò alla smilitarizzazione, sindacalizzazione e apertura all'arruolamento femminile della Polizia di Stato, con la legge n. 121 del 1981, in anni duri e complessi quali quelli in cui lo Stato e le istituzioni dovettero affrontare e superare l'emergenza del terrorismo. Per quanto riguarda la legge Mammì sull'emittenza radiotelevisiva, occorre ricordare che il progetto iniziale di riforma rimase nei cassetti e che la versione votata dal Parlamento, che avrebbe assunto il suo nome, non aveva un firmatario e fu il risultato di un compromesso al ribasso tra le diverse forze politiche. Come è noto, fu determinante l'impulso del PSI di Craxi, il quale impose il voto di fiducia al Governo. Il provvedimento disciplinava il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, incaricandosi di fotografare *de iure* il monopolio di fatto dell'imprenditore Silvio Berlusconi in ambito televisivo, nella fondamentale sfera della raccolta pubblicitaria e stabilendo che le sue tre reti private, in un regime di duopolio con la RAI, avrebbero dovuto dotarsi di appositi telegiornali.

si dimisero il 27 luglio 1990 dal Governo, ma furono avvicendati senza colpo ferire dal presidente del Consiglio Andreotti. Questa è la data di inizio della carambola italiana 1990-1993, in cui si definirono assetti di potere, conflitti di interesse e alleanze politiche di lunga durata in ambito interno ed internazionale. Mammì ha attraversato con disciplina, onore e una buona dose di pungente ironia la stagione della cosiddetta Prima Repubblica, quella del protagonismo politico e civile dei partiti. Pur non avendolo conosciuto di persona, immaginiamo che abbia guardato con distacco Non a caso, si ritirò dalla vita politica attiva, in silenzio, dopo l'implosione di quel sistema dovuto alla crisi di Tangentopoli

desidero porgere le nostre condoglianze ai familiari tutti, a quanti gli hanno voluto bene e in particolare a sua figlia Alessandra. signori del Governo, colleghe e colleghi, se dopo venticinque anni dalla conclusione dell'attività parlamentare Oscar Mammì viene ricordato in quest'Aula con le parole di rispetto e di considerazione che gli sono state rivolte da tutti i colleghi che mi hanno preceduto, evidentemente

di politico che ha svolto l'attività parlamentare attraversando venti anni di storia, dal 1972 al 1992 (ben cinque legislature), di uomo di Governo, con incarichi di Sottosegretario prima e di Ministro dopo.

caratteristica in particolare, quella della coerenza, che emerge in modo puntuale e preciso, indipendentemente dalle valutazioni di merito che si possono fare sull'efficacia dell'azione politica

credo che emerga con assoluta chiarezza la grande coerenza che nel tempo Oscar Mammì ha mantenuto nel rapportarsi al patrimonio di valori di laicismo del Partito Repubblicano. Fu un uomo senz'altro colto, di grande cultura, ma dotato anche di grande arguzia politica, di grande senso di ironia e di lealtà, più propenso e incline all'attività di mediazione e di composizione tra posizioni differenti che non a percorrere la strada dello scontro. Credo che la sua attività abbia trovato, dopo l'impegno politico, un riscontro singolare e significativo anche in quella *fiction* televisiva alla quale si è fatto riferimento, allorquando, vestendo i panni dell'innominato, partecipò alla *fiction* «Walter e Giada» ispirata a «I promessi sposi». Egli stesso sostenne, in un'intervista, che uno che fa politica o è un buon attore oppure non ce la fa e lui fece anche l'attore. Fu anche significativo il senso che diede all'interpretazione del ruolo dell'innominato. Egli disse cioè che la rappresentazione del potere aveva caratteristiche sempre uguali nel tempo: è sempre quello, ciò che cambia è la democrazia. Mammì disse: nel tempo, si lavorava prima per costruire il consenso; oggi invece si cerca di capire dove va il consenso e poi ci si regola di conseguenza. Ecco la coerenza, credo la lezione migliore, che rappresenta il lascito di Oscar Mammì, con cui diamo forza

grato e solidale alla sua famiglia. Signor Presidente, sarò brevissimo, non perché la figura di Oscar Mammì non meriti di parlare a lungo della sua storia politica e personale, ma perché ho poco da aggiungere rispetto a quanto è stato detto dai dai colleghi che mi hanno preceduto. Non ho avuto la fortuna di conoscere personalmente Oscar Mammì, quindi non ho aneddoti da raccontare, tranne uno che ho rilevato leggendo la sua biografia e che mi ha colpito, una delle sue interviste, che evidenzia la sua capacità

in occasione della sua apparizione televisiva. «L'Innominato è la rappresentazione del potere, che ha caratteristiche uguali nel tempo. Il potere è sempre quello, è cambiata certo, e in peggio, la nostra democrazia: un tempo si lavorava per costruire il consenso, ora si cerca di sapere dove va il vento e lo si segue». Una sferzata a una politica miope, incapace di guardare al futuro e di costruire una classe dirigente degna di questo nome, in quanto arroccata nella salvaguardia dell'esistente. Mammì ha rappresentato una lunga, memorabile, orgogliosa parte della storia del repubblicanesimo italiano. Fu sempre convinto che la crisi italiana fosse superabile unicamente attraverso un impegno politico e non certo attraverso soluzioni istituzionali o giudiziarie. Auspichiamo che queste parole e quello che abbiamo sentito in quest'Aula non cadano nel vuoto e che vi sia uno sforzo costante nell'impegno politico attivo delle nuove generazioni. Noi di Alternativa Popolare, anche nel rispetto delle storie di appartenenza di molti di noi alle tradizioni repubblicane e, in passato, al Partito Repubblicano, ci uniamo al ricordo di Oscar Mammì e siamo vicini alla famiglia e ai parenti tutti.

Ovvio il ricordo di alcuni passaggi legislativi importanti, non solo legati a una legge che ha segnato un momento fondamentale della vita parlamentare e democratica, ma anche del suo amore per la vita politica. Voglio ricordarlo, anche da romano, come protagonista della vita politica romana; anche questo tratto Non posso non aggiungere anche un ricordo personale, di quando, nel 2002, Mammì era lontano dal Parlamento da tempo e avemmo un dibattito, promosso da Bruno Vespa, nel momento in cui mi toccò innovare nel campo delle televisioni la legislazione

Credo che il mondo sia andato avanti e sia stato ulteriormente innovato. Per me è stato dunque un riferimento, nella discussione e nel confronto, nei processi di modernizzazione dell'informazione e del sistema radiotelevisivo

finanze*. Signor Presidente, desidero soltanto aggiungere che il Governo si associa al ricordo di Oscar Mammì e al cordoglio per la sua scomparsa.

Signor Presidente, userò meno del tempo a disposizione perché vogliamo arrivare presto alla votazione di queste mozioni. Si è perso fin troppo tempo. Innanzitutto, vorremmo esprimere un giudizio su quanto avvenuto questa mattina, perché riteniamo molto grave che il Partito Democratico e la maggioranza abbiano tentato di minimizzare la gravità della vicenda Consip. Qui non stiamo parlando di «strumentalizzazioni politiche», come è stato maldestramente affermato nella discussione di questa mattina, ma di gravi casi di corruzione. Non è ancora chiaro, naturalmente, il livello di coinvolgimento delle figure istituzionali accusate, ma i fatti vanno accertati. E non ci piace l'atteggiamento del Governo e della maggioranza: quando le indagini riguardano i propri sodali il PD è garantista; quando coinvolgono gli avversari politici diventa giustizialista. Ormai ci siamo abituati. Questo atteggiamento non ci stupisce più e, fortunatamente, anche i cittadini hanno capito il vostro gioco e la vostra ipocrisia. Ma veniamo alla vicenda Consip. Consip gestisce gare d'appalto milionarie per la pubblica amministrazione. Quando sono stati assegnati questi ruoli si sapeva che avrebbe mosso grandi interessi. Sarebbero stati necessari controlli eccezionali e grande attenzione. Invece le indagini della magistratura, immancabilmente, hanno evidenziato gravi casi di corruzione. Abbiamo assistito all'arresto dell'imprenditore Alfredo Romeo, che avrebbe corrotto funzionari Consip e avrebbe promesso denaro a Tiziano Renzi, padre dell'allora Presidente del Consiglio e dell'attuale segretario del Partito Democratico. Abbiamo assistito all'avviso di garanzia nei confronti di un Ministro, Luca Lotti. Non un Ministro qualsiasi. Per altri Ministri, per episodi molto meno gravi sono arrivate le dimissioni. Per Lotti no. È uno del Giglio Magico. Uno dei più discussi collaboratori di Matteo Renzi. A lui tutto è permesso e perdonato. Accusato di aver informato dirigenti Consip dell'esistenza delle indagini in corso è ancora al suo posto. È ancora un potente Ministro della Repubblica. L'amministratore delegato di Consip, Luigi Marroni, avrebbe confermato alla magistratura la veridicità di tali circostanze, ed è forse per questo che se ne deve andare. Per mesi si è chiesto di trattare la vicenda Consip in Parlamento. La maggioranza lo ha consentito solo dopo le dimissioni dei componenti del consiglio e Marialaura Ferrigno. Ci chiediamo quindi se queste siano state circostanze casuali, dimissioni spontanee, fatti non correlati. Onestamente, è difficile pensarlo. In ogni caso, vorremmo rispondere al presidente Zanda e al Partito Democratico, che parlano di questione superata e di caso risolto, che noi non siamo assolutamente d'accordo: la decadenza del consiglio di amministrazione di Consip non risolve nulla. Non risolve gli scandali, le responsabilità penali e neppure quelle politiche. Non volevate questo dibattito. Volevate insabbiare tutto. Ma non ci riuscirete, nonostante la vostra ipocrisia e la vostra arroganza! È ormai chiaro che il Governo, il PD di amministrazione di Consip e soprattutto del suo amministratore delegato solo perché ha parlato, ha collaborato con la magistratura; perché è colui che con le sue dichiarazioni ha messo nei guai Luca Lotti, l'amico di Renzi. Voi non volete realmente mettere ordine in Consip. Stiamo assistendo ad un regolamento di conti all'interno della maggioranza. Renzi e il PD vogliono solo fare piazza pulita di uomini coinvolti in indagini molto gravi e pericolose, che hanno toccato persino la famiglia del capo, i suoi amici, i suoi sodali. In tutta questa vicenda c'entra poco la politica. In questa vicenda sembrano essere coinvolti i vertici di un sistema di potere che vogliono difendersi dalle indagini, spostare l'attenzione dell'opinione pubblica, trovare un unico capro espiatorio, rimuovere gli ostacoli, rimuovere scomodi testimoni. Noi della Lega Nord non ci stiamo; non accettiamo questa ignobile farsa. Noi pretendiamo la verità; la pretendono i cittadini. Vogliamo sapere in definitiva se siamo stati governati da uomini perbene o da un comitato d'affari. *(Applausi

e di una parte della maggioranza: un'ostinazione, peraltro illogica, visto che sono anche decaduti, in gran parte, i presupposti, a voler discutere a tutti i costi di mozioni non tanto per capire davvero cos'è accaduto in Consip, come qualcuno ha detto, ma - questa è la verità - per puntare ancora una volta il dito nei confronti del Governo, e in particolar modo nei confronti del ministro Lotti. Accuse basate solo su illazioni che non hanno alcun fondamento. Questo a me appare ancora più paradossale e illogico perché sulla vicenda Consip credo ci sia ben altro da dire, ben altro su cui discutere. Mi riferisco all'indagine sul depistaggio: all'indagine sul depistaggio: un'indagine basata non su supposizioni, ma su intercettazioni chiare, direi inequivocabili. Tutto questo ai danni dell'allora presidente del Consiglio Matteo Renzi. Questo è, a mio avviso, un fatto gravissimo, inaccettabile, che dovrebbe sollevare un coro unanime di sdegno da parte di tutte le forze politiche; un coro unanime di sdegno e di richiesta di chiarimento, questa Un fatto così grave perché riguarda tutti noi; riguarda la democrazia di questo Paese. Colleghi, non so voi, ma io sono letteralmente stanca di questi vent'anni di scontro ideologico che ha paralizzato il nostro Paese, che lo ha portato all'immobilismo più totale, che lo ha portato alla crisi sociale e politica in cui oggi si trova. Per questo, mi appello qui oggi a tutti, a un maggiore senso di responsabilità perché sono certa di una cosa, che vi è una lezione che avremmo dovuto imparare già da tempo

PLI))*. Signora Presidente, non credo che la discussione di oggi sia paradossale. Anzi mi permetto di rilevare, rispetto alla collega che mi ha preceduto, che almeno la mozione a prima firma

ma cercava di disincagliare le pessime abitudini del Parlamento, e di questo ramo del Parlamento, quell'inutile, grottesco e giacobino strumento della mozione individuale di sfiducia nei confronti del singolo Ministro. Questa è una vicenda abbastanza lunga, lunga, da quando fu introdotto nel nostro Regolamento questo strumento. Un professore di diritto parlamentare, che poi è diventato senatore e nostro collega, di una certa autorevolezza, non dell'opposizione di centrodestra, ma del Partito Democratico (parlo del professor Andrea Manzella), lo definì un'inutile *gadget* istituzionale, nel senso che, dal punto di vista della politica costituzionale, il voto di fiducia è un nesso che lega l'istituzione Governo all'istituzione Parlamento

è una fregnaccia. D'altra parte, essa è nel nostro Regolamento. Insieme a quei 72 colleghi della mozione Augello di qualche mese fa, cercammo di discutere in Senato di altra materia rispetto a quella sulla quale il Senato era stato sollecitato. In quell'occasione il presidente Grasso, assai meno colloquiale e disponibile di stamattina, fu molto arcigno e disse che di ciò,

che sarebbe stato molto evasivo da parte di un'Assemblea parlamentare. Il comportamento del singolo Ministro e le sue deleghe, fra l'altro in materia di sport, presso la Presidenza del Consiglio non c'entrano assolutamente niente. Il problema - scusate se è poco, attendo con molta passione l'intervento di un rappresentante del Governo come Morando - La Consip è stata inserita nel nostro ordinamento mi pare di capire sentendo la diatriba statutaria - un pochino "a capocchia", perché in quella che avrebbe dovuto essere, ai vertici dello Stato repubblicano, la centrale degli acquisti della pubblica amministrazione ha prevalso la politica "politicante". Sono un garantista, anzi psicologicamente sono un innocentista prescindo perciò dai profili di diritto e di procedura penale. Tra i personaggi che si agitano attorno a questa vicenda vi

che arrivano a Confindustria dopo essere attentamente passati per una vicenda politica. Il personaggio proviene dalla cosiddetta "destra comunista napoletana", cioè il mondo del PCI-PDS.

nel senso che devo dire di aver firmato la mozione Augello perché nel marzo di quest'anno nessuno poneva il problema di un chiarimento indispensabile da parte di chi aveva il compito di nominare e anche rimuovere i membri del consiglio di amministrazione e la presidenza della Consip. In quella mozione erano anticipati argomenti che poi, ho apprezzato, sono stati inseriti nella mozione a prima firma del senatore Zanda. Per cui oggi,

E allora è necessario che le future nomine dei membri del consiglio di amministrazione della Consip siano più accurate e confacenti al ruolo terzo che compete a un'istituzione qual è la Consip.

e ufficiali di polizia giudiziaria che hanno sicuramente svolto attività non confacenti al ruolo, o quanto meno la cui coerenza con l'obbligo della funzione deve essere verificata dall'autorità giudiziaria. Noi dobbiamo fare scelte politiche. Mi sia allora consentita una brevissima considerazione sulle società, nazionali e anche regionali, che devono sovraintendere la funzione dell'istituzione appaltante. Non sono convinto che stia andando tutto bene. Lo dico ai rappresentanti del Governo e richiamo anche l'attenzione di certa magistratura su alcune società regionali. Voglio fare un nome per tutte: la So.Re.Sa, la società

di queste istituzioni, che - ribadisco - devono avere un ruolo assolutamente terzo e non possono essere disponibili a preconfezionare fotografie che sono già leggibili per i futuri destinatari delle forniture.

un'azione chiarificatrice da parte di altri, dobbiamo invocarla anche per quanto riguarda quelle realtà che derivano dalla responsabilità nostra e delle maggioranze che sosteniamo.

di valutazioni che risiedono nell'opportunità dei singoli o delle forze politiche o coalizioni cui appartengono. Rileviamo semplicemente

derivano dai presunti risparmi che l'attività di Consip può portare nel panorama della spesa pubblica; risparmi che non solo non si sono verificati,

gli appalti di Consip diventano sempre più grandi e sappiamo benissimo che con la grandezza degli appalti aumentano gli appetiti e i margini per fare cose che non si dovrebbero.

Questo al Paese interessa relativamente (o almeno dovrebbe interessare relativamente), ma serve invece una riflessione puntuale e profonda sul ruolo di Consip e, ad esempio sugli effetti che questo continua delegare a Consip competenze e funzioni ha, di riflesso, sull'attività degli enti locali, molto spesso costretti ad inseguire le gare di Consip e a pagare le forniture ad un prezzo superiore rispetto a quello che potrebbero trovare sui mercati locali di riferimento.

ogni volta sempre maggiori compiti a Consip. Proprio questo è l'argomento che dovrebbe essere in discussione. Consip dovrebbe essere più un'autorità regolatrice dei prezzi di spesa della pubblica amministrazione, che non un'autorità di vera e propria attribuzione attribuzione di appalti in materia di grandissime spese a livello nazionale. Quindi, se dal dibattito dovesse uscire questa riflessione, allora certamente faremo cosa utile per il Paese, ma se ci limitiamo alle considerazioni

Presidente, vengo subito alla formulazione dei pareri, perché sarà attraverso il parere che si capirà il punto di vista e la valutazione del Governo sulla questione al nostro esame.

Essa infatti - questa è la ragione del parere favorevole - prende esplicitamente e positivamente atto delle novità intervenute nel corso di questi ultimi giorni

rigorosamente la legislazione e la regolazione vigente. Non si tratta infatti solo di leggi, ma anche di regolamenti e direttive che riguardano le nomine nelle società partecipate, controllate, possedute dal Ministero dell'economia e delle finanze.

alla luce di un indirizzo esplicito: prende atto, come è stato dichiarato di recente anche dal Ministro dell'economia, dell'esigenza di tutelare la funzione assolutamente cruciale di Consip per migliorare l'efficienza della spesa pubblica e per realizzare risparmi significativi sul versante dell'acquisizione di beni e servizi e, positivamente valutando ciò che è intervenuto, impegna il Governo a fare nomine che siano coerenti con il rilievo che Consip ha in questo momento.

Sulla parte delle premesse e delle motivazioni il parere del Governo è contrario. Sulla parte dispositiva, quella degli impegni al Governo, quest'ultimo è favorevole al primo e al terzo impegno, non è invece favorevole - e ne spiego rapidamente le ragioni - al secondo impegno.

potrà eventualmente essere presa in considerazione l'esigenza di intervenire con sospensioni di gare. Ma noi non possiamo prima impegnarci a sospendere gare in forza di una dichiarazione giornalistica di qualcuno per poi impegnarci a verificare attraverso un'inchiesta amministrativa se effettivamente queste pressioni, a proposito di questa o quella gara, ci siano state e abbiano manifestato i loro effetti. Per questa ragione, se si proponenti fossero d'accordo con la proposta che sto avanzando, ci dovrebbe essere soltanto una piccola modifica, meramente formale ma conseguente all'ipotesi di

PLI))*. Signor Presidente, colleghi, signori del Governo, prima di dichiarare il voto del mio Gruppo, comunque andrà la votazione consentitemi di esprimere sincera soddisfazione e lasciatemi ringraziare il senatore Andrea Augello e i 73 colleghi che hanno sottoscritto la mozione che ha dato vita a questo dibattito. Cento giorni fa, quando la nostra mozione è stata presentata, in discussione nel caso Consip c'erano rapporti patologici tra affari e politica e un'inchiesta compromessa da una clamorosa fuga di notizie. Nel frattempo si è aggiunto un terzo dato: la presunta alterazione di alcuni elementi relativi a un altro filone d'indagine. Per quanto ci riguarda, noi non abbiamo mai pensato che il giudizio penale dovesse entrare in questa Assemblea. Ma abbiamo respinto con altrettanta fermezza l'idea per la quale la non interferenza nel lavoro della magistratura potesse rappresentare un alibi per sottrarsi anche al giudizio sui comportamenti politico-istituzionali. se non tocca a noi stabilire chi tra Luca Lotti e Luigi Marroni dice la verità e chi mente, certamente tocca a noi affermare che il Governo, nel momento in cui sceglie di schierarsi, non può schierarsi contemporaneamente a difesa dell'uno e dell'altro, dell'accusato e dell'accusatore, del sedicente calunniato e del presunto calunniatore. Ancora. Lasciare la giustizia ai tribunali non significa non prendere atto che taluni comportamenti pubblicamente rivendicati dall'amministratore delegato della Consip integrano una manifesta violazione del codice etico. Non significa non rilevare come il titolare del Ministero che della Consip è socio unico abbia cambiato idea con la stessa disinvoltura con la quale si cambia il guardaroba con i primi caldi. Ci sono voluti cento giorni perché di tutto ciò si potesse discutere in questa ancora nelle ultime ore e giorni sono successe cose rilevanti: il PD ha deciso di unirsi con una propria mozione alla richiesta di azzeramento dei vertici della società. Nel farlo, non è comunque restato neutrale nello scontro giudiziario tra Lotti e Marroni, ma ha preso posizione per il primo. Questo è il punto che differenzia la nostra posizione da quella del PD. Nel frattempo, il Ministro che aveva sempre difeso la permanenza in carica dell'amministratore delegato, si è adoperato per far cadere l'intero consiglio di amministrazione, ottenendo le dimissioni di due consiglieri su tre, ma non quelle di Marroni. il presidente di Consip Luigi Ferrara, che nelle stesse ore è stato indagato per false dichiarazioni al pubblico ministero in merito a quella stessa fuga di notizie che era stata il terreno di scontro tra Marroni e Lotti. hanno rafforzato le ragioni a sostegno della necessità di un dibattito parlamentare. Un dibattito che si sarebbe potuto affrontare cento giorni fa, ma che comunque cento giorni dopo ha finalmente messo fine a una situazione di palese e insostenibile contraddizione. Per quel che ci riguarda, signor Presidente, rivendichiamo la linearità di una posizione istituzionalmente rigorosa, ma che nulla ha mai concesso al giustizialismo. Rivendichiamo come una vittoria nostra e dei colleghi che ci hanno affiancato in questa lunga battaglia l'azzeramento di una dirigenza inadeguata a guidare la più importante stazione appaltante del nostro Paese. Rivendichiamo come una vittoria il fatto che questo dibattito si sia svolto, e che si sia svolto con approccio civile e secondo una dinamica fisiologica tra Parlamento e Governo, laddove il Parlamento ha evidenziato le incongruenze del Governo e l'ha richiamato ai suoi compiti. Rivendichiamo, inoltre, di aver posto tutti i protagonisti della vicenda, a cominciare dall'amministratore delegato della Consip, nelle migliori condizioni, anche formali, per dire tutto ciò che sanno. Rivendichiamo, infine, di aver reso evidente agli occhi del Paese chi è che vuole chiarezza e chi invece fa di tutto per occultare la verità. Nel ringraziare nuovamente il Senato per la prova di maturità, annuncio per ciò il voto favorevole del Gruppo Federazione della libertà

Signor Presidente, quanto è avvenuto oggi nell'Aula del Senato ha veramente del surreale: siamo partiti, questa mattina, con la richiesta da parte del Partito Democratico di rinviare - o meglio sarebbe dire insabbiare - questo dibattito.

che viene chiamato in causa per questioni che in altri tempi avrebbero prodotto l'interevento della Corte marziale, quando c'è una condizione per la quale viene chiamato in causa

fatto diventare il nostro. Leggo direttamente dall'articolo di giornale: «È insomma la cronaca di una deposizione suicida quella di Ferrara. In cui il presidente dimissionario di Consip si mette nella condizione di chi o ha mentito prima (ai pm di Napoli) o sta mentendo dopo (ai pm di Roma). E che, per giunta, nei toni sconclusionati che ad un certo punto avrebbe assunto - al punto dal rendere impossibile persino la verbalizzazione sintetica delle sue dichiarazioni e consigliare l'immediata interruzione dell'atto con la contestazione delle "false o reticenti informazioni al pubblico ministero" - suggerisce l'idea di un uomo prigioniero di pressioni insostenibili o comunque incomponibili».

se siamo giunti al dibattito non è per la volontà divina di fare chiarezza, ma perché c'è un'opposizione come la nostra che non vuole fare sconti alle nefandezze che questo Governo ormai da troppo tempo sta facendo. Voi oggi avete individuato un capro espiatorio il paradosso è che l'amministratore delegato di Consip va a riferire ai magistrati e oggi viene messo sul banco degli imputati da parte del Governo e del PD con la mozione in cui sostanzialmente si individua in lui il responsabile della situazione, lasciando totalmente intonse e non citando le responsabilità del ministro e allora sottosegretario Lotti. Voi oggi potete fare tranquillamente buon viso a cattivo gioco facendo finta di niente, ma dovete essere consapevoli che il Paese non ne può più di questo vostro modo di fare da amici del quartierino, anzi da amici della loggia del quartierino. Questa, infatti, è la situazione con cui vi state caratterizzando al Governo: state facendo gli amici della loggia che fanno gli affari al Governo e questa è una cosa che non vi potete permettere e che, soprattutto, non

verità, a deporre. Chiediamo quindi come potete conciliare l'incoerenza di rimanere in un Governo che respinge la mozione con la quale

Mi viene poi da interrogarmi sulla coerenza dell'altra parte della maggioranza: penso al partito di Alfano, che forse più di MDP ha trovato un particolare equilibrio di coerenza. Come farà a confrontarsi

Noi non voteremo niente che faccia pressioni nei confronti di chi è andato a rendere testimonianza davanti alla giustizia. Siate voi a prendervi questa responsabilità, perché ormai il fetore di quello che state facendo non lo si sente solo in quest'Aula, ma lo si legge tutti i giorni sui giornali.

il tempo è un grande attore e trova sempre un'ottima soluzione per il finale. L'unico finale che possiamo augurare a questo Governo è che la legislatura si concluda immediatamente con un voto contrario e che metta finalmente il Governo davanti alle proprie responsabilità. È iscritta a parlare la senatrice Repetti. il tratto distintivo della vicenda Consip è, come ha ricordato nel suo intervento di questa mattina il senatore Gotor, la commistione tra affari, politica e istituzioni, che si evince dalle reti strette, i legami amicali, i favori e le pressioni che ci vengono raccontate. In questo contesto, concentrare l'attenzione sui soli vertici Consip è, secondo noi, limitativo, insufficiente e, per certi versi, fuorviante. La nostra mozione, pur amputata nel dispositivo, conserva un tratto che la distingue da tutte le altre: nella nostra mozione, infatti, e solo nella nostra, si afferma come imprescindibile l'indissolubilità del legame tra le vicende del ministro per lo sport Luca Lotti e quelle dell'amministratore delegato di Consip, dottor Luigi Marroni. Per questo, voteremo a favore della nostra mozione, mentre esprimeremo un voto contrario sulle altre. il Gruppo per le Autonomie-PSI-MAIE ritiene che sarebbe stato opportuno il rinvio del dibattito parlamentare in merito alle mozioni sul caso Consip. Le dimissioni giunte al Ministero di due dei tre consiglieri d'amministrazione della Consip comporta, come noto, ai sensi dello statuto, le dimissioni dell'intero organo; dimissioni delle quali il ministro Padoan ha informato l'Assemblea

Luca Lotti, condividiamo il giudizio di improponibilità, per estraneità di materia, espresso dal presidente Grasso. Abbiamo sempre auspicato e sostenuto una lettura equilibrata e ispirata ad indispensabili princìpi di cautela del caso Consip, mentre, al contrario, dobbiamo purtroppo constatare come l'esigenza, del tutto condivisibile, di piena trasparenza sia stata manipolata da alcuni per ragioni del tutto strumentali, cercando in modo improprio e infondato di chiamare in causa responsabilità di Governo. Vista l'importanza del sistema Consip, riteniamo invece prioritario che il Governo proceda in tempi celeri al rinnovo dei vertici, scegliendo tra personalità

ci pone di fronte alla necessità di tutelare, con un'azione di bilanciamento ed equilibrata valutazione, rilevanti interessi pubblici. La Consip, quale società per azioni del Ministero dell'economia, suo azionista unico, opera secondo i suoi indirizzi strategici al servizio esclusivo della pubblica amministrazione. I risultati in questa direzione, come sottolineato in alcune mozioni oggi in discussione, sono certamente positivi. Senza entrare di nuovo nei dati di dettaglio, basti ricordare che, nell'ultimo triennio, i risparmi cumulati dall'area pubblica grazie all'azione della Consip sono stimati in oltre 11 miliardi di euro. Ma perché, allora, alcune mozioni richiedono il ricambio dei vertici dell'azienda? Ovviamente la risposta è da ricercare nei fatti, anche penalmente rilevanti, che hanno coinvolto da una parte soggetti partecipanti alle gare bandite da Consip e dall'altra i suoi massimi dirigenti, oltre ad alcuni esponenti politici. Il complesso delle situazioni venute in rilievo getta un'ombra pesante sull'opportunità di consentire di continuare la gestione dell'azienda alle personalità finora in carica. Da una parte non vorrei addentrarmi nei dettagli dell'inchiesta, articolata in diversi filoni, in diversi filoni, composta da contestazioni diversificate a differenti soggetti e complicata anche dal punto di vista tecnico. In questo senso dobbiamo ribadire la necessità di rispettare il lavoro della magistratura, rinnovando piena fiducia agli inquirenti. Siamo certi che sapranno condurre le operazioni in modo da ricostruire in modo preciso e coerente le dinamiche dei fatti, anche correggendo alcune distorsioni che pure si sono verificate, come tutti sappiamo. In questo contesto, il ruolo assunto dai vertici Consip rispetto ad alcune interazioni e, in alcuni casi, interferenze esterne da soggetti a vario titolo interessati all'espletamento delle procedure per l'aggiudicazione dei lotti di cui si compone la macro gara d'appalto (in particolare la gara del cosiddetto *facility management*, FM4) sono divenute di pubblico dominio, rispondente ai doveri d'ufficio e alle precauzioni dovute. A prescindere dalle contestazioni che attengono all'inchiesta penale, in questa sede siamo chiamati a valutare agli articoli 54, 97 e 98, la Carta ci dice che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione e adempiono alle funzioni pubbliche loro affidate con disciplina

L'impegno della mozione a prima firma Zanda mira proprio a restituire il più alto grado di credibilità alle azioni dei soggetti e alle attività istituzionali della società, prendendo atto delle dimissioni dei rappresentanti del MEF dal consiglio di amministrazione Consip, da cui discende la necessità giuridica di rinnovare l'intero consiglio. L'unica possibilità per restituire dignità politica e fiducia nelle future politiche della Consip è quella di dare, con coraggio, un segno di completa discontinuità con il passato, nell'attesa che le singole responsabilità penali vengano accertate e, se del caso, sanzionate dalla magistratura.

politico di fondo che dovrebbe interessare tutti quanti noi e su cui il Governo, a maggior ragione, avrebbe dovuto pronunciarsi e dare alcune risposte riguarda l'elemento che ha

molto pesante e pericolosa tra affari e politica e su come sono stati scelti i vertici della Consip: in base a quale richieste e in base a quali influenze. Oggi ho parlato della politica di politica di una certa Provincia che a un certo punto ha preso il potere nel nostro Paese e che ha cominciato a piazzare i suoi uomini un po' dappertutto

ha prodotto un meccanismo a catena, che concentrava sulla Consip molta attenzione, visto il volume degli affari, e le questioni ci sono state. È vero che la faccenda dovrà essere accertata,

viene accusato di avere messo sull'allerta lo stesso amministratore delegato sull'indagine in corso. Un quadro, dal nostro punto di vista, desolante.

dice innanzi tutto che la Consip nasce per un processo di razionalizzazione della spesa pubblica, delle risorse, per condurre tutte le varie centrali di acquisti ad un'unica centrale sulle amministrazioni. Ebbene, oggi scopriamo - e qui c'è un problema molto grave - un sistema di concentramento anche nel modo di gestire gli appalti molto preoccupante. Su questo non vi è alcuna risposta né sull'indagine amministrativa né rispetto al futuro, e si spera che le nomine future siano fatte secondo le procedure previste.

Gruppo dico che, per quanto ci riguarda, guardiamo alla sostanza; guardiamo esattamente quello che è scritto nelle mozioni. Invito tutti una volta per tutte, soprattutto su questioni e dibattiti come questi,

alcune scelte di altri colleghi, ma ognuno ovviamente è libero. Per quanto ci riguarda, ci atterremo solo ed esclusivamente a quanto c'è scritto. Non possiamo certamente votare la mozione

C'è scritto: «impegna il Governo a procedere in tempi celeri e solleciti al rinnovo dei vertici della Consip». Siccome lo statuto della Consip dice che, decaduti due su tre, ma anche solamente uno, risulta decaduto il consiglio di amministrazione, non ho capito che cosa impegneremmo la Consip o il Governo a fare. Lo si impegna a fare una cosa che deve già fare? Ma io capisco perché voi scrivete una cosa di questo tipo. È da mesi che dite che l'amministratore delegato Marroni se ne deve andare. siccome Marroni non se ne va e non volete prendervene voi la responsabilità, volete che sia il Parlamento a dire al Governo di farlo. In questo modo l'italiano deficiente - è evidente che l'italiano, secondo voi, è un deficiente - non se ne accorge. Peccato che l'italiano non sia deficiente e che di questo se ne sia accorto. E comunque noi stiamo dicendo al caro italiano di svegliarsi. Ma andiamo avanti. Secondo voi - è scritto nel dispositivo - la Consip è una cosa fantastica e svolge attività di assistenza e supporto agli acquisti della pubblica amministrazione. Fa questo. Nel corso degli anni ha fatto belle cose e ha avuto grandi competenze. C'è scritto questo. Quindi cosa c'entra? Questa è la domanda. Noi stiamo parlando d'altro. Stiamo parlando non della sostituzione dei vertici, ma di questo, perché è successo qualcos'altro. Vogliamo fare un elenco di quanto è successo, giusto per dire le due cosette che sono capitate? Per esempio, è successo che il presidente della Consip ha fatto una dichiarazione, che poi ha ritrattato - una deposizione poi ritrattata - nella quale ha tirato in ballo nientemeno che il comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Ma di questo voi non fate menzione nella mozione. Non è niente, no? Ma non basta. È stato tirato in ballo il comandante dell'Arma della Toscana - mica della Micronesia, ma della Toscana - che avrebbe fatto una rivelazione di segreto d'ufficio. È andato a dire

Ma di cosa stiamo parlando, del niente? A chi stiamo raccontando questa balla? Quindi, ricapitoliamo: ci sono di mezzo il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che è indagato per rivelazione di segreto d'ufficio; il comandante territoriale della Regione Toscana; un imprenditore che voleva entrare nella torta di 2,7 miliardi; il padre dell'ex Presidente del Consiglio; il braccio destro dell'ex Presidente del Consiglio (Lotti). Secondo voi, però, questo non è il problema. Anzi, bisognava aspettare il 27 del mese per poter dire che è tutto risolto, che il consiglio di amministrazione è stato azzerato e va tutto bene. Ma è uno scherzo? Se è uno scherzo, non è divertente. Qua non ride nessuno. nessuno. La verità è che quella che voi portate avanti è un'operazione di puro insabbiamento: la testa è sotto la sabbia e tutto il resto del corpo è fuori. Ma voi sperate veramente che l'inchiesta si possa chiudere una volta che avete tolto di mezzo il cappello

Ma, soprattutto, vale la pena di fare tutta questa manfrina per proteggere l'ex Presidente del Consiglio? Alla fine davanti a lui avete alzato i muri e scaricato tutto quello che potete scaricare. Renzi non si tocca. Non si tocca lui. Non si tocca suo padre. Non si tocca Lotti, che è il Ministro dello sport. Ci siamo inventati pure il Ministro dello sport. "Ma de che? Stamo nel fascismo?" Ci siamo inventati anche questo. Ma Renzi non si deve toccare. Renzi, che ha portato questa Nazione al fondo, non deve essere toccato. Allora noi diciamo, dopo il patetico tentativo di stamattina di cercare di non far discutere le mozioni, che le mozioni finte come la vostra non devono neanche essere prese in considerazione. Invece le altre hanno motivo di essere prese in considerazione, compresa la riformulazione che è stata richiesta al senatore Augello e che noi riteniamo corretta. Quello che è giusto è giusto. Ma, siccome quello che è giusto è giusto, ha ragione anche la Lega, quando dice che vi dovete assumere la responsabilità di quanto andrete a combinare. Se voi rimuovete impropriamente il consiglio di amministrazione, ve ne assumete la responsabilità. Non può poi diventare colpa di qualcun altro. Ogni responsabilità, anche politica, va assunta. Noi ci siamo veramente stufati del vostro metodo. Ma non basta, perché bisogna aggiungere anche altro. C'era di mezzo

al ministro Lotti, il Gruppo di Forza Italia sostenne, in coerenza con la linea di non sostenere per principio le mozioni di sfiducia individuali, che non si sarebbe per l'appunto votato quell'atto parlamentare.

poi in realtà molto italiano e molto vicino alle italiche tradizioni, quelle un po' consuetudinarie e non molto nobili: il babbo, il papà, quell'altro, i parenti, gli amici, Marroni e i sodali nominati a destra e manca. Non voglio riaprire quella discussione che poi sui giornali si rinnova ancora: la telefonata del babbo alla Ministra e al Presidente del Consiglio (uno dei due babbi, quello famoso in materia bancaria) poi il babbo di Rignano. Insomma, mi pare che questa vicenda, politicamente, abbia già dimostrato al gruppo di potere che l'arroganza non paga. E lo si è visto al *referendum*; lo si è visto nel percorso delle riforme e lo si è visto persino a Rignano,

Il risultato politico è stato già raggiunto e ha fatto bene il senatore Augello ad accettare le riformulazioni proposte dal Governo. Quindi, il Gruppo di Forza Italia voterà quella mozione che ha sostenuto, condiviso e che ha raggiunto il risultato.

Ed è anche una soddisfazione poter denunciare questa vicenda. Quindi la conseguenza si è già avuta. In tutta la vicenda di intercettazioni, vere o presunte, vorrei

al Ministro e agli altri ci penseranno gli elettori. Noi crediamo nella democrazia salvifica. Quindi, il risultato politico è stato raggiunto. In conclusione, si è tentato

sia nata in un quadro molto diverso da quello determinato ora dalle dimissioni del consiglio di amministrazione di Consip. Quello della messa in discussione dei vertici di Consip era ed è il senso di molte delle mozioni presentate oggi. Per questo motivo, non le voteremo,

del quadro nuovo che si è determinato e guardano ai compiti che la politica, il Parlamento e il Governo hanno di fronte sulla vicenda Consip. È nostra volontà impegnare il Governo a rinnovare rapidamente il consiglio di amministrazione di Consip dopo le dimissioni dei consiglieri. Sollecitiamo inoltre un rafforzamento del *management* che produca un rafforzamento dell'attività e della funzione di Consip per centralizzare gli acquisti, controllare

intervenuti. È ovviamente legittimo, anzi doveroso esplicitare le opinioni diverse, ma trovo meno comprensibile l'idea di risollevare questioni su cui il Senato si è

si corra a invocare processi sommari, a pronunciare invettive o promulgare sentenze. Non è serio nei confronti del Parlamento usare quest'Assemblea e la discussione sulla Consip (sul suo funzionamento e non sull'inchiesta) per alimentare sospetti, fare insinuazioni, costruire dietrologie Non vedo la volontà in alcuni di capire che cosa è successo davvero, in una vicenda integrata, in cui - ricordo - le inchieste sono due. Vedo solo la volontà di continuare a ripetere tesi precostituite. A noi interessa fare chiarezza su ciò che è accaduto. Ad altri interessa solo avere qualcosa da strumentalizzare, per gettare discredito sull'avversario politico. Interventi come quello che ho sentito questa mattina come quelli della Lega non fanno bene alla politica, al Parlamento e agli occhi dei cittadini, ai quali si dice che la politica è una palude, in cui tutto si spiega e tutto avviene per volontà di oscuri poteri, comitati d'affari e forze occulte. E, soprattutto, gli argomenti usati screditano - e mi dispiace - chi li usa, perché si preferisce cercare un facile consenso, assecondando l'idea purtroppo diffusa tra i cittadini che tutta la politica è marcia, e sposare una tesi precostituita, piuttosto che fare la fatica di cercare la soluzione dei problemi, la trasparenza e la verità, per capire che cosa è successo davvero. Questo interessa ai cittadini. Questo interessa al PD e su questo continueremo a impegnarci. Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione.

sulla deliberazione sul parere espresso dalla 1a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti

Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento e le chiedo di dirimere una questione che era stata posta dal senatore Calderoli, ma anche dal nostro Gruppo, la settimana scorsa.

entro cinque giorni dalla richiesta, i presupposti di costituzionalità in Aula. I cinque giorni sono passati e oggi siamo al sesto giorno. Di fatto, ancora è in piedi un decreto che doveva essere votato. Il Regolamento è chiaro: entro cinque giorni il Presidente del Senato mette ai voti

a quale parte del Regolamento ci si appiglierà questa volta per il solito *escamotage.* E ci dica a chi possiamo appellarci per poter chiedere una revisione della decisione che la Presidenza sappiamo già che prenderà, calpestando i diritti di questo Parlamento.

Presidente, se lei procede con l'esame dei presupposti di costituzionalità e urgenza, di cui parla il senatore Crimi, noi ci troviamo assolutamente d'accordo. Se così fosse, andiamo avanti, perché ritengo assolutamente legittime le richieste del senatore Crimi.

è stata portata all'attenzione dell'Assemblea e il diritto parlamentare ha delle regole sulla giustiziabilità che sono codificate dalla nostra Costituzione, per cui alcune norme sono

Richiedo un chiarimento ai sensi dell'articolo 78, comma 3. Lei ha detto un'inesattezza, perché c'è scritto che il Presidente del Senato o sottopone il parere entro cinque giorni al voto dell'Assemblea. Il Presidente del Senato ha sottoposto il parere entro i cinque giorni la settimana scorsa ed essendoci,

secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente, per il disegno di legge n. 2856: «Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale». Ricordo che

e cito tutti i precedenti che vanno nel seguente senso: esame dei presupposti, manca il numero legale e l'esame è rinviato all'11 gennaio 1995. Presupposti conclusi.

da una parte una difficoltà, perché purtroppo la prassi che lei ricordava - quei tre precedenti - esiste veramente. Io non capisco come tutte le volte la Presidenza possa andare alla ricerca di un precedente che faccia comodo in quel momento, dimenticandosi del Regolamento.

non è la fattispecie di mancanza del numero legale quella che si è verificata. E, quindi, quel precedente viene invocato a sproposito. Le faccio notare, però, che c'è stato un atto di prepotenza. Ascolti me, per favore. PRESIDENTE. La ascolto, io sono *multitasking*: riesco ad ascoltare e a leggere

Signora Presidente, anche dopo una verifica sommaria con gli altri Gruppi, credo che potrebbe essere opportuno iniziare la trattazione di un provvedimento che sta a cuore

io ritengo che ci sia una prassi nella storia delle assemblee parlamentari in prossimità di una competizione elettorale. Come noi sappiamo, domenica ci sono i ballottaggi,

Senatore Mancuso, non ho capito cosa ha detto alla fine, se è favorevole o contrario

dal 15 giugno scorso al prossimo 7 luglio sono in corso a New York i lavori della Commissione che sta trattando l'argomento delle armi nucleari.

Noi abbiamo intenzione di presentare una questione pregiudiziale e una sospensiva: vorrei sapere se le dobbiamo presentare subito dopo la relazione del senatore Lumia - lo

Presidente, colleghi, la riforma al testo unico antimafia giunge finalmente all'approvazione dell'Assemblea. Non è stato facile: il cammino legislativo è stato lungo, complesso, anche con problemi di copertura finanziaria di non facile soluzione, ma adesso ci siamo. Il testo, ricordo a tutti i colleghi, è già stato approvato alla Camera; adesso, migliorato e completato dal lavoro della Commissione giustizia del Senato, ci consente di fare quel salto di qualità nella lotta alle mafie così atteso da anni, forse anche da troppi. Insieme con il collega relatore, senatore Pagliari, affronteremo due parti complessive di questa vasta riforma. La riforma è composta da 36 articoli suddivisi in sette capi. Sostanzialmente, la prima parte affronta la riforma e la disciplina delle misure di prevenzione personali e patrimoniali; la seconda parte affronta l'altro vasto argomento della riforma dell'Agenzia che interviene e gestisce i beni confiscati. Per quanto riguarda la prima parte, l'articolo 1 interviene sull'articolo 4 del codice antimafia inserendo tra i possibili destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, anche fuori dal caso di concorso o di favoreggiamento, gli indiziati di prestare assistenza agli associati per quanto riguarda le organizzazioni a delinquere e mafiose (articolo 418 del codice penale). Anche questa è un'innovazione importante, attesa da anni, che completa il novero dei soggetti da aggredire sul versante della lotta alla mafia. C'è stato anche un importante inserimento fatto dalla Camera: quello di annoverare tra i soggetti da colpire con le misure di prevenzione, soprattutto patrimoniale, gli indiziati di una serie di reati contro la pubblica amministrazione. Rispetto al testo licenziato dalla Camera dei deputati, la Commissione ha ulteriormente esteso l'ambito soggettivo di applicazione, ricomprendendovi anche coloro che sono indiziati di uno dei delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo, già richiamati dal comma 3-*quater* dell'articolo 51 del codice di procedura penale, ma sistematizzati meglio con la riforma e con gli interventi della nostra Commissione giustizia. Sono stati poi previsti anche i soggetti coinvolti nei delitti di atti persecutori (l'articolo 612-*bis*, sempre del codice di procedura penale), che tutti annoveriamo tra i reati di *stalking*. Anche questa è una innovazione molto importante e attesa, in quanto quel tipo di reato va affrontato soprattutto in fase di prevenzione, visto che, tra l'altro, esso è strutturato con una serie di condotte ripetute che ricadono proprio nell'ambito dell'abitualità e della pericolosità sociale del soggetto. Sappiamo tutti che spesso questo tipo di reato apre la strada al femminicidio. Pertanto, è stato importante questa proposta, proposta, accolta ed inserita all'interno della riforma proprio in Commissione giustizia. Per i soggetti che consumano i reati di truffa aggravata

attentato, quasi una strage, nei confronti del presidente di quel Parco, Giuseppe Antoci, e degli uomini della sua scorta), abbiamo inserito, nel corpo e nel novero di questa riforma, altre misure, che vanno a colpire

Tanto è vero che in questa riforma, proprio in Commissione giustizia, abbiamo alzato, per quanto riguarda proprio questo tipo di reato, la pena:

proprio quell'accesso alla gestione e all'affitto dei terreni che, cari colleghi, addirittura supera per redditività il traffico così opulento di cocaina. Ecco perché abbiamo voluto, da questo punto di vista, prevedere che il famoso protocollo del Parco dei Nebrodi, noto proprio come protocollo Antoci, diventasse anche norma, in modo che lo Stato possa autorizzare questa sperimentazione, farla propria e la faccia diventare un sistema ordinato di intervento per colpire le ricchezze che si stanno accumulando, non solo in Sicilia, ma su tutto il territorio nazionale. Prevediamo, inoltre, la possibilità che gli enti parco, sia regionali che nazionali, diventino, insieme agli altri enti istituzionali locali, destinatari di gestione a fini sociali e produttivi proprio di beni sequestrati e confiscati alla mafia. La Commissione ha inoltre modificato l'articolo 4, comma 1, lettera *f)*, del codice antimafia, prevedendo che le misure di prevenzione personali si applichino anche a coloro che compiono atti esecutivi (a (a legislazione vigente unicamente atti preparatori) diretti alla ricostituzione del partito fascista. Cari colleghi, l'articolo 2 reca modifiche al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali. La disposizione interviene, in primo luogo, sull'articolo 5 del codice antimafia, prevedendo che il procuratore della Repubblica del circondario, nelle specifiche ipotesi in cui la titolarità della proposta di misure di prevenzione personale spetti anche a questi, adotti la proposta previo coordinamento con il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto; e che la proposta di misura debba essere depositata, non più presso il tribunale del capoluogo della Provincia in cui dimora il soggetto proposto, bensì presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi speciali per le misure di prevenzione del tribunale del capoluogo del distretto nel territorio del quale la persona dimora. Sezioni e collegi istituiti dal successivo articolo 31 del disegno di legge. Anche questa è una misura che qualifica il codice antimafia perché crea delle sezioni specializzate, in grado di avere quindi un giudice ben preparato capace di aggredire il cuore del potere mafioso,

sviluppata la pericolosissima mafia dei Casalesi), la Commissione ha previsto che tale proposta debba essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi specializzati in materia di misure di prevenzione ivi istituiti, nel caso in cui la persona dimori nel corrispondente circondario. L'articolo in esame modifica, poi, l'articolo 6 del codice antimafia, prevedendo che il divieto di soggiorno possa essere applicato anche in relazione

Sono apportate, inoltre, numerose modifiche all'articolo 7 del codice antimafia che disciplina il procedimento applicativo delle misure personali. Sinteticamente, si prevede: che i trenta giorni entro cui il tribunale deve pronunciarsi decorrono dal deposito della proposta;

del giudice; la possibilità, in casi particolari, di sentire con il collegamento a distanza anche soggetti informati sui fatti. Sempre in Commissione giustizia qui al Senato è stato aggiunto il comma 4*-bis* all'articolo 7 del codice antimafia, con il quale si prevede che il tribunale, dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, ammette le prove rilevanti, escludendo quelle vietate dalla legge (o superflue, ovviamente). È stato poi aggiunto al comma 5 un periodo nel quale si prevede un'ulteriore causa di rinvio dell'udienza per l'applicazione delle misure di prevenzione, quando, però, sussiste un legittimo Il disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera, aggiunge, sempre all'articolo 7 del codice antimafia, nuovi commi che recano un'articolata regolamentazione delle questioni concernenti la competenza territoriale, volta a dirimere alcune questioni lungamente dibattute a livello giurisprudenziale. In base alla nuova disciplina, tali questioni devono essere eccepite a pena di decadenza alla prima udienza, e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti, e il tribunale le decide immediatamente. immediatamente. Possono essere rilevate di ufficio naturalmente, con la decisione, di primo grado. Se ritiene la propria incompetenza, il tribunale la dichiara con decreto ordinando la restituzione degli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente (anche se è diverso l'organo proponente). La declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. La stessa disciplina trova applicazione anche nel caso in cui la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore legittimati ai sensi dell'articolo 5 del codice antimafia. Quando il tribunale accoglie l'eccezione d'incompetenza, il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se entro venti giorni dal deposito del provvedimento il tribunale competente (se investito dal pubblico ministero competente che ha ricevuto gli atti) non dispone il sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali, oggi dovute solo per il giudizio di Cassazione. Sempre con riguardo all'articolo 7 del codice antimafia, la disposizione reca una puntuale disciplina in tema di termini di deposito del decreto del tribunale. Il decreto deve essere infatti depositato entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza. Quando la stesura delle motivazioni è particolarmente complessa, il tribunale, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni. Il termine può essere ulteriormente prorogato di centottanta giorni ai sensi dell'articolo 154 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. L'articolo 2 modifica infine l'articolo 8 del codice antimafia, prevedendo che il decreto del tribunale possa contenere, tra le prescrizioni, il divieto di soggiorno in una o più Regioni e che la decisione del tribunale debba essere comunicata anche al difensore del proposto. L'articolo 3, avente ad oggetto la disciplina delle impugnazioni delle misure di prevenzione personali, interviene sull'articolo 10 del codice antimafia, permettendo la proposizione del ricorso in appello e in Cassazione anche al difensore dell'interessato (attualmente il solo legittimato). L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 14 del codice antimafia, relativo a decorrenza e cessazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Si prevede in primo luogo che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. Il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare, con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi. Oltre a prevedere che l'esecuzione della sorveglianza speciale resti sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena, la nuova disciplina stabilisce che la verifica della pericolosità avvenga ad opera del tribunale (anche d'ufficio), dopo la cessazione della detenzione che si è protratta per almeno due anni, attraverso un articolato procedimento. A tale riguardo, in Commissione giustizia è stato approvato un emendamento che precisa che la suddetta verifica della persistenza della pericolosità sociale avvenga sentito il pubblico ministero che ha esercitato le relative funzioni nel corso della trattazione camerale, assumendo le necessarie informazioni, oltre che presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza, anche presso gli organi di polizia giudiziaria. Se la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione; se invece persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato. È opportuno osservare come le modifiche testé illustrate mirino a disciplinare gli effetti della sentenza della Consulta n. 291 del 2013, con cui è stata dichiarata l'illegittimità l'illegittimità costituzionale degli articoli 12 della legge n. 1423 del 1956 e 15 del codice antimafia, nella parte «in cui non prevedono che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura». Il capo II del provvedimento (composto da diversi articoli, dal 5 al 12) modifica la disciplina delle misure di prevenzione patrimoniali. L'articolo 5 interviene sulla disciplina relativa al procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, esplicitando, con riguardo alla titolarità della proposta, i poteri di coordinamento del procuratore della Repubblica distrettuale e circondariale

al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto sono attribuite anche al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona, previo coordinamento con il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto. Nei medesimi casi, nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione, le funzioni di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. La disposizione interviene poi in materia di sequestro (articolo 20 del codice antimafia) stabilendo che, oltre al sequestro di valori ingiustificati ritenuti probabile frutto di attività illecita, il decreto del tribunale può disporre anche l'amministrazione giudiziaria di aziende, nonché di beni strumentali all'esercizio delle relative attività economiche. In questo modo il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie è esteso *ex lege* a tutti i beni aziendali: un'innovazione importante, tra le tante che da anni ci vengono richieste dagli operatori che agiscono contro la mafia in questo delicato settore e che richiede anche una *technicality* che sia in grado di allargare l'ambito di intervento di sequestro e di confisca. Per quanto riguarda l'esecuzione del sequestro (articolo 21 del codice antimafia), la disposizione del disegno di legge in esame prevede che alla materiale apprensione dei beni sequestrati e all'immissione dell'amministratore giudiziario nel loro possesso provvede la polizia giudiziaria (anziché l'ufficiale giudiziario). Capirete naturalmente anche la portata di questa innovazione. Naturalmente l'assistenza di quest'ultimo rimane solo eventuale («ove opportuno»). In Commissione giustizia è stato rivisto il testo dell'articolo 21 del codice antimafia - rispetto alla formulazione recata dal disegno di legge approvato dalla Camera - sostituendo il comma 2 nel senso di prevedere che il giudice delegato alla procedura, ai sensi dell'articolo 35, comma 1 (anziché il tribunale), sentito l'amministratore giudiziario, valutate le circostanze, ordina lo sgombero degli immobili occupati senza titolo, ovvero sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro mediante l'ausilio della forza pubblica. Sono stati poi soppressi i commi da 2-*bis* a 2-*quinques* dell'articolo 7 introdotti dalla Camera che regolavano le modalità di sgombero degli immobili da parte del tribunale. L'articolo 5 del disegno di legge interviene poi in materia di sequestro d'urgenza, stabilendo che il decreto che dispone la misura di prevenzione perde efficacia se non è convalidato dal tribunale entro trenta giorni. giorni. L'articolo 5 del disegno di legge in oggetto dispone che il proposto non possa giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia frutto di evasione fiscale:

di cui adesso tratterà il relatore Pagliari, finalmente comporta trasparenza, efficienza ed energie organizzative e professionali, per fare in modo che anche i beni confiscati diventino una risorsa e non più un problema nella lotta alle mafie. Chiedo alla Presidenza Signora Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito di premettere una breve riflessione all'illustrazione del provvedimento. Considero questo incarico di relatore il più significativo della mia esperienza parlamentare. Pur nella consapevolezza della modestia del mio ruolo, contribuire a costruire la legislazione contro la mafia e combattere la criminalità organizzata nell'esercizio della funzione parlamentare è un onore e una grande gratificazione. Non posso proprio per questo omettere di ricordare le vittime della mafia, della 'ndrangheta e della camorra, da quelle più oscure a quelle più famose, da quelle uccise e vittime di violenza a quelle vittime della criminalità organizzata nella vita quotidiana e apparentemente normale di tutti giorni, da quelle che subiscono la criminalità organizzata nelle terre di tradizione a quelle che subiscono la prepotenza e le angherie nelle terre di attuale infiltrazione, a cominciare dalla mia Regione, l'Emilia Romagna, e dalla mia città, Parma. Men che meno voglio dimenticare coloro che combattono quotidianamente la criminalità, dall'associazione Libera agli amministratori pubblici, ai tanti cittadini che senza pubblicità sono quotidiani e indifesi combattenti contro questo tumore. Mi si lasci fare, infine, un'ultima considerazione. Con la novella il codice antimafia si applicherà anche ai responsabili di reati contro la pubblica amministrazione, corruzione in testa. Come non cogliere in questo precetto una denuncia decisa e un richiamo a combattere anche la mafia di fatto, quella determinata dai contesti dominati dal malaffare, dal clientelismo e dall'illegalità, quella che crea lo Stato nello Stato nei contesti più diversi e insospettabili, assoggettando le istituzioni agli interessi di pochi e precludendo le funzioni pubbliche a tutela di tutti e la fruibilità delle istituzioni a coloro che non si piegano. La mafia si combatte anche contrapponendosi a questi fenomeni. Il capo III del provvedimento modifica la disciplina in tema di amministrazione, gestione e destinazione di beni sequestrati e confiscati. L'articolo 13 del disegno di legge interviene sulle norme del codice antimafia che definiscono i criteri per la scelta degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati e regolano gli adempimenti connessi alla cessazione del loro incarico. La disposizione prevede, in primo luogo, che qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, il tribunale può nominare più amministratori eventualmente stabilendo se essi debbono operare congiuntamente o disgiuntamente. A un successivo decreto ministeriale è demandata la definizione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari, nonché l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo di incarichi. La norma, poi, oltre a prevedere che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, reca puntuali cause ostative all'assunzione di tale incarico. In Commissione giustizia è stato introdotto un comma aggiuntivo 35 del codice antimafia, secondo cui, fermo restando quanto previsto per il sequestro di aziende di straordinario interesse socioeconomico, l'amministratore giudiziario giudiziario possa essere nominato anche tra il personale dell'Agenzia di cui all'articolo 113-*bis*. In tal caso, l'amministratore giudiziario dipendente dall'Agenzia per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto a emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, a eccezione di un rimborso spese. Ancora, la disposizione riconosce all'amministratore giudiziario la facoltà di organizzare, su autorizzazione del giudice delegato, un proprio ufficio di coadiuzione. L'articolo 13 del disegno di legge introduce poi nel codice antimafia un nuovo articolo 35-*bis*, relativo alla responsabilità nella gestione e ai controlli della pubblica amministrazione. Ancora, l'articolo 13 modifica l'articolo 36 del codice antimafia sulla relazione dell'amministratore giudiziario. L'articolo 14 modifica la disciplina della gestione dei beni sequestrati e confiscati, con particolare riferimento alla gestione delle aziende. Più nel dettaglio, il disegno di legge interviene sull'articolo 40 del codice antimafia con modifiche volte a consentire l'utilizzo dei beni immobili sequestrati fin dalla fase dell'esecuzione, con l'ausilio dell'agenzia nazionale. Si introduce, all'uopo, un'articolata disciplina diretta a guidare l'attività del tribunale e del giudice delegato, attraverso il recepimento di alcune prassi virtuose. In estrema sintesi, nel caso di immobili dati in locazione o comodato con data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione dei contratti alla scadenza naturale. Invece, nel caso di immobili liberi ovvero liberati, l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può in via prioritaria, anche su proposta su proposta dell'agenzia, concedere in comodato i beni ai soggetti cui il bene può essere destinato o assegnato dopo la confisca definitiva, con cessazione alla data della confisca definitiva, ovvero locare o concedere in comodato i beni, prevedendo la cessazione nei casi da ultimo esposti e, comunque, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva. Per i beni mobili l'articolo prevede norme più stringenti per evitare inutili custodie, imponendo la vendita se i beni non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie e la distruzione o demolizione se privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili. La disposizione reca una disciplina più compiuta in materia di reclamo degli atti dell'amministratore giudiziario posti in essere in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato. L'articolo 14 riscrive, poi, l'articolo 41 del codice antimafia, disciplinando analiticamente i contenuti della relazione che l'amministratore giudiziario deve presentare entro tre mesi dalla nomina; in particolare egli dovrà descrivere le concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, allegando un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, dalla relazione di un professionista, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo. Nella proposta di prosecuzione l'amministratore dovrà altresì censire i creditori dell'azienda e i lavoratori impiegati. Si consente all'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, di affittare l'azienda o un ramo d'azienda, o concederla in comodato. Da ultimo la disposizione contempla, in assenza di concrete possibilità di prosecuzione dell'attività, modalità semplificate di liquidazione o cessazione dell'impresa. L'articolo 15 del disegno di legge inserisce nel codice antimafia il quale introduce gli strumenti finanziari di sostegno e valorizzazione delle aziende sequestrate necessari per la legalizzazione delle attività non irreversibilmente inquinate dai capitali o dai metodi "illeciti".

L'articolo 16 inserisce nel codice antimafia il nuovo articolo 41-*ter* con il quale si istituiscono presso le prefetture dei tavoli permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, ai quali sono chiamati a partecipare, oltre ad un rappresentante dell'Agenzia La funzione dei tavoli permanenti è di favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende, per favorire la continuità produttiva e la conseguente salvaguardia dell'occupazione. I tavoli esprimono un parere non vincolante sulle proposte dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia. L'articolo 16 introduce poi nel codice antimafia l'ulteriore articolo 41-*quater*, il quale dispone che l'amministratore giudiziario, dopo aver sentito il competente tavolo permanente, e previa autorizzazione del giudice delegato, possa avvalersi del supporto tecnico, gratuito,

l'amministratore dovrà presentare una volta divenuta irrevocabile la confisca - e alla gestione dei beni confiscati da parte dell'Agenzia. L'articolo 18 interviene sulla destinazione dei beni confiscati, modificando alcune disposizioni del codice antimafia. In particolare inserisce nel codice l'articolo 45-*bis*, con il quale è disciplinata la liberazione e lo sgombero dell'immobile e delle aziende; modifica l'articolo 46 confermando la possibile restituzione per equivalente, in caso di restituzione di beni confiscati; interviene sull'articolo 47 del codice, relativo al procedimento di destinazione, disponendo che, se si attivano le procedure a salvaguardia dei terzi o dei creditori, l'Agenzia deve adottare il provvedimento di destinazione entro novanta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento dei crediti. In relazione alla destinazione dei beni e delle somme, disciplinata dall'articolo 48 l'articolo 18 del disegno di legge prevede che la vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie sia consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda o di beni immobili e che la vendita delle partecipazioni societarie possa essere effettuata solo con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti e la destinazione del bene agli enti territoriali per finalità economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali. La disposizione, oltre ad introdurre più puntuali misure dirette ad assicurare la pubblicità da parte degli enti territoriali dei beni a loro destinati, così come delle assegnazioni, prevede l'assegnazione, a titolo gratuito, direttamente da parte dell'Agenzia agli enti o alle associazioni sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri che devono essere stabiliti dal consiglio direttivo dell'Agenzia. In Commissione giustizia è stato introdotto il comma 15-*ter* dell'articolo 48 del codice che le previsioni sulla destinazione dei beni immobili di cui al comma 3 si applicano anche gli immobili confiscati già facenti parte del patrimonio aziendale di società le cui partecipazioni sociali siano state confiscate in via totalitaria o comunque tali da assicurare il controllo della società. L'Agenzia, con delibera del consiglio direttivo può dichiarare, tuttavia, la natura aziendale dei predetti immobili, ordinando al conservatore dei registri immobiliari la cancellazione di tutte le trascrizioni pregiudizievoli al fine di assicurare l'intestazione del bene in capo alla medesima società. L'articolo 19 modifica l'articolo 51 del codice antimafia, sul regime fiscale dei beni sequestrati per specificare che, se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha inizio, il reddito derivante dal bene è determinato dall'amministratore giudiziario in via provvisoria, ai soli fini fiscali. Il capo IV del disegno di legge modifica la disciplina del codice antimafia relativa alla tutela dei terzi ed ai rapporti con le procedure concorsuali. In particolare, l'articolo 20 modifica i seguenti articoli per variare le condizioni in presenza delle quali i diritti di credito dei terzi non vengono pregiudicati; l'articolo 53, per specificare che dalle somme per la soddisfazione dei crediti per titolo anteriore al sequestro, della quale si fa carico lo Stato nel limite cento del valore di stima del bene sequestrato, devono essere sottratte le spese del procedimento e di amministrazione dei beni; l'articolo 55, che dispone la sospensione delle procedure esecutive già pendenti al momento del sequestro e l'estinzione delle stesse in caso di confisca definitiva; l'articolo 56, relativo ai rapporti pendenti al momento del sequestro, che stabilisce che se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in se il contratto relativo all'azienda sequestrata o al bene in sequestro deve essere ancora eseguito, l'esecuzione resta sospesa fintanto che l'amministratore giudiziario non dichiara di subentrare. L'articolo 20 del disegno di legge inserisce inoltre nel codice antimafia l'articolo 54-*bis* (pagamento di debiti anteriori al sequestro), per il quale il giudice delegato può autorizzare l'amministratore giudiziario a pagare o rinegoziare debiti pregressi relativi a rapporti commerciali necessari per la prosecuzione dell'attività. L'articolo 21 detta disposizioni relative all'accertamento dei diritti dei terzi. Il disegno di legge modifica in primo luogo l'articolo 57, sull'elenco e la verifica dei crediti, per specificare che nell'elenco dei creditori devono essere inseriti anche coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia e per ridurre da novanta a sessanta giorni il termine perentorio che il giudice assegna ai creditori per il deposito delle istanze di accertamento dei crediti. La disposizione modifica poi l'articolo 58, sulle domande di ammissione del credito, disciplinando più rigorosamente la presentazione delle istanze tardive, prevedendo il coinvolgimento dell'amministratore giudiziario nel procedimento. Oltre a limitate modifiche alla verifica dei crediti e alla composizione dello stato passivo di cui all'articolo 59 del codice antimafia, il disegno di legge interviene sulla fase della vendita e liquidazione dei beni (articolo 60 del codice antimafia) nonché sulla fase del progetto e del successivo piano di pagamento dei crediti che inizia dopo l'irrevocabilità del provvedimento di confisca, divenendo di competenza dell'Agenzia. L'articolo 22 disciplina i rapporti con le procedure concorsuali, modificando gli articoli 63 e 64 del codice Si interviene in materia di dichiarazione di fallimento successiva al sequestro prevedendo una più precisa disciplina della verifica dei crediti operata dal giudice delegato alla prevenzione con riferimento ai beni assoggettati a sequestro o confisca, esclusi dalla massa attiva fallimentare, e dal giudice delegato al fallimento per i restanti anche dopo la revoca del sequestro. La disposizione stabilisce inoltre che, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, l'amministratore giudiziario può, previa autorizzazione del tribunale: presentare al tribunale fallimentare domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti della legge fallimentare; presentare domanda per l'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* legge fallimentare; predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera *d)*, della legge fallimentare, finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva e il mantenimento dei livelli occupazionali. Nessuna modifica è invece apportata alla vigente disciplina nella parte in cui non consente al tribunale di proporre la richiesta di fallimento. L'articolo 22 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 64 (sequestro successivo alla dichiarazione di fallimento) attribuendo al giudice delegato della prevenzione le verifiche dei crediti con riferimento ai beni assoggettati a sequestro, anche se già verificati dal giudice delegato al fallimento.

altre sanzioni penali; l'articolo 25, recante modifica dell'articolo 83 del codice antimafia relativamente all'ambito di applicazione della documentazione antimafia. L'articolo 26 modifica l'articolo 84 del codice antimafia attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo infiltrativo anche al coinvolgimento in procedimenti penali per il reato di caporalato. Il capo V del provvedimento interviene sulle disposizioni del codice antimafia relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo come sede principale

In Commissione giustizia è stata poi riportata l'Agenzia sotto la vigilanza del Ministro dell'interno, come attualmente previsto dal codice antimafia, e si sono accentuate le competenze consultive del Comitato consultivo

ed introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 113-*ter*), che prevede il conferimento di incarichi speciali a personale con qualifica dirigenziale o equiparata, fino al limite massimo di dieci unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, Forze di polizia ed enti pubblici economici, comandato o distaccato o collocato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni istituzionali II capo VI contiene modifiche al codice penale, alle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e alle leggi speciali, nonché varie deleghe al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità

Signora Presidente, mi faccio, in quest'Aula questa sera, portatore delle istanze e delle preoccupazioni dei dipendenti - e delle loro famiglie - dell'azienda Tecnomessapia, un vero e proprio fiore all'occhiello della Puglia, e non solo, che negli anni ha raggiunto traguardi importantissimi nell'ambito della qualità produttiva del settore aeronautico. Tecnomessapia ha aumentato la sua forza lavoro, passando da 80 a più di 400 dipendenti, lavorando in appalto per società controllate da Finmeccanica. Quest'ultima, nel 2015, per un processo di internalizzazione, ha proceduto a fare un vero e proprio travaso di competenze presso altri stabilimenti, avvalendosi del personale di Tecnomessapia che di fatto ha proceduto a trasferire il proprio *know how* specifico ad operatori di altre aziende. Una volta completato l'affiancamento, però, il personale Tecnomessapia è stato dichiarato in esubero. Il 30 giugno prossimo si procederà al licenziamento degli ultimi 175 dipendenti.

Chiedo quindi, attraverso di lei, signora Presidente, che il ministro De Vincenti, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, provveda ad anticipare la data, prevista per metà luglio, di convocazione del tavolo sulla crisi occupazionale, che insiste in modo molto preoccupante sul tessuto economico e sociale di Brindisi e della Puglia

Solo attraverso una sinergia tra Regione e Governo nazionale si potrà infatti disinnescare il rischio ormai concreto di un vero e proprio *shock* occupazionale per il territorio brindisino, dove gli indici socioeconomici sono già attestati su livelli di grande preoccupazione. inoltre consentita un'ulteriore precisazione. Spetta *in primis* al Governo garantire interventi urgenti e coraggiosi per contrastare la crisi occupazionale in atto in molti territori.

Signora Presidente, desidero sollecitare la risposta a varie interrogazioni inerenti il mio territorio, la Lombardia. La prima riguarda la vergognosa situazione di Seregno, in cui diversi esponenti della Lega Nord si sono dimessi dai loro incarichi a motivo della pesantezza della situazione, che vede interessi della 'ndrangheta orbitare in città in modo molto marcato, come ho dimostrato negli atti ispettivi

«Preferirei esser governato dalla mafia piuttosto che dallo Stato italiano. La mafia al Sud almeno, qualche servizio lo dà, lo Stato italiano usa i miei soldi per pagare Gad Lerner, Michele Santoro, quelli della RAI». Successivamente avrebbe aggiunto: «La mafia, se io mi difendo dal ladro, non viene a mettermi in galera (...) Le tasse che lo Stato italiano mi mette sono come il pizzo della mafia al Sud, con la differenza che lo Stato italiano non smette mai di mettermele».